esteri*. Signor Presidente, signore senatrici e signori senatori, il 12 giugno ho riferito alla Camera sugli eventi in Turchia e sono lieta di fornire oggi un aggiornamento al Senato. La linea che l'Italia ha tenuto è stata ed è centrata su due cardini. Il primo: abbiamo insistentemente rivolto al Governo turco - l'ho fatto personalmente anche in un recente colloquio telefonico con il ministro degli esteri Davutoglu un forte appello alla moderazione e alla ricerca di soluzioni condivise: sono le espressioni, proprio nei momenti critici, di una democrazia partecipativa e matura. Reazioni sproporzionate non sono mai negli interessi né di un popolo al quale ci sentiamo molto vicini, il popolo turco, né del Governo di un Paese che voglia definirsi quale democrazia compiuta. al secondo cardine: abbiamo sottolineato nei colloqui con i nostri *partner* europei, anche recentemente nel Consiglio affari esteri di lunedì, che l'Unione europea non può cedere alla reazione istintiva di irrigidirsi, di chiudersi di fronte ai fatti che hanno travagliato la Turchia. Può non essere intuitivo; ma se adottiamo, come è doveroso da parte dei Governi, un atteggiamento ragionato e strategico, la realtà è che dobbiamo invece tenere aperto il canale del dialogo. Perderemmo, altrimenti, qualunque possibilità di influenza. Il processo dì adesione all'Unione europea ha sempre dimostrato di essere una potente leva di impulso alle riforme democratiche dei Paesi candidati e al rafforzamento delle loro istituzioni. Non è un caso che da quando l'obiettivo dell'integrazione europea si è affievolito le riforme in Turchia abbiano subito un rallentamento. Se vuole influenzare il percorso democratico e riformista della Turchia, l'Europa non può e non deve congelare i negoziati. Per quanto riguarda le decisioni prese al Consiglio affari generali di martedì scorso hanno segnato un passo importante a favore di questa impostazione italiana. La formula di compromesso individuata - con una decisione di principio favorevole all'apertura del capitolo 22 il rinvio ad una successiva discussione in autunno per definire la data della Conferenza intergovernativa - è stata accolta in modo positivo anche da parte turca (me lo ha confermato il ministro Davutoglu martedì Lo stesso primo ministro Erdogan ha espresso apprezzamento per questa soluzione. Il dialogo resta dunque aperto, come ritenevamo giusto. Si è evitato il muro contro muro. Questo è un importante passo avanti accettato anche da alcuni dei Paesi europei inizialmente contrari all'apertura del capitolo 22. Ma lo ripeto: è una decisione strategica, nell'interesse del popolo turco e dell'Unione europea. Se la decisione di Lussemburgo va quindi salutata con favore, molto dipenderà - naturalmente - dagli ulteriori sviluppi in Turchia, che seguiremo con attenzione. Il nostro obiettivo è chiaro: riuscire progressivamente ad integrare la Turchia in Europa, e una Turchia che si dimostri pienamente democratica. Emarginare o spingere Ankara verso altri poli di attrazione non sarebbe né negli interessi di un'Europa che ha nel fronte mediterraneo un fronte vulnerabile, né negli interessi di un popolo, quello turco, che ancora aspira - per lo meno in percentuali rilevanti - ad un ancoraggio europeo. europeo. Sui fatti e sulla prima fase della protesta ho già riferito la settimana scorsa. Il Governo italiano continuerà a sensibilizzare quello turco perché, come richiesto anche da mozioni presentate qui in Senato, sia fatta luce su quanto avvenuto, inclusi gli asseriti casi di violenza su donne, che ad oggi non hanno tuttavia trovato conferma ufficiale. La Farnesina - con l'unità di crisi, la nostra ambasciata ad Ankara e i nostri consolati a Istanbul e Smirne - ha seguito sin dall'inizio gli avvenimenti, prestando particolare attenzione alla presenza e alla tutela di cittadini italiani. A essere coinvolto negli scontri, come sapete, è stato anche il fotografo italiano Daniele Stefanini, che è stato posto in stato di fermo mentre faceva delle foto nella zona di piazza L'intervento della nostra ambasciata ad Ankara e del nostro consolato generale a Istanbul ha consentito il rilascio, il giorno successivo, del signor Stefanini, che ha fatto immediatamente rientro in Italia. Nel frattempo, il vice presidente dell'AKP, Celik, ha annunciato che il futuro di Gezi Park sarà deciso con un *referendum*. L'ipotesi di una consultazione locale per decidere le sorti del parco era stata già ventilata dal vice primo ministro Arinç, come forse sapete. Onorevoli senatrici e senatori, mi avete sentito ripetere più volte che piazza Taksim non è piazza Tahrir. La Turchia ha radici democratiche, i partiti al Governo e il Primo Ministro sono stati liberamente eletti e per tre volte hanno ricevuto un chiaro mandato popolare. Ma l'iniziativa dei cittadini indica che una parte di loro non si riconosce nell'evoluzione più recente del partito AKP. Sarà anche una minoranza nel Paese, come è stato detto, ma, come riconosciuto anche da autorevoli esponenti politici e osservatori turchi, la democrazia non significa solo vincere le elezioni. Significa anche sapere ascoltare la voce dei cittadini e tutelare le opinioni delle diverse componenti della società, ammettendo che possano essere espresse in modo pacifico. La tutela delle minoranze, infatti, è l'autentico *test* di maturità democratica: per tutti i Paesi, inclusa la Turchia. In questi anni l'Italia ha sempre guardato con fiducia al modello turco, nella convinzione che fosse capace di coniugare islam e democrazia. È forse illusorio pensare che il solo successo economico - e non c'è dubbio che il Governo Erdogan abbia prodotto notevoli risultati i economici - non generasse tensioni sociali. Come ha scritto in modo efficace Samuel Huntington, nelle società dove si sperimentano trasformazioni rapide che producono un aumento rapido della classe media, le domande che derivano dalla società aumentano a velocità più sostenuta delle capacità dei Governi a soddisfarle. In sintesi, da una parte Ankara ha riscosso significativi risultati, come da ultimo importanti misure di apertura alla componente curda. Quest'ultima, non a caso, è stata per lo più assente dalle manifestazioni di piazza. D'altra parte, esistono segnali di malessere nella società, come il disagio crescente per un insufficiente rispetto della libertà di espressione. I *Progress report* dell'Unione europea fanno stato di questo quadro, fatto di luci e ombre. E per esprimere una valutazione obiettiva occorre tener conto di questo insieme composito, senza passare da un eccesso all'altro. Se fino a qualche settimana fa la Turchia era indicata come un modello da seguire, ora non dobbiamo cedere a un pessimismo eccessivo. L'Italia ha gli strumenti culturali e sociali per comprendere meglio di altri Paesi la complessità delle società, e della società turca, perché anche il nostro Paese è un microcosmo in cui negli anni, storicamente, si sono verificate, su scala diversa e con le dovute distinzioni, tensioni causate dal contrasto tra aspirazioni liberali e risposte di chiusura. L'ancoraggio europeo ha permesso all'Italia di superare tante crisi e sacche di arretratezza, assicurandoci maggiore libertà, e sarebbe sbagliato negare oggi questa stessa possibilità al popolo turco. Tenere in vita i negoziati è tenere in vita questa possibilità. L'esito finale dipenderà dai progressi concreti che verranno compiuti sui vari capitoli negoziali. Eancora non sono stati aperti - ci torno tra un momento - i capitoli cruciali che riguardano diritti umani, libertà e giustizia (in particolare i capitoli 23 e 24). Vedremo nei prossimi mesi. Infine, l'Europa. Onorevoli senatrici e senatori, come detto all'inizio, la decisione raggiunta a Lussemburgo sull'apertura del capitolo 22 è un segnale positivo, ma dobbiamo dirci onestamente qualche verità. I negoziati erano in una fase di stallo da tempo, e per altre ragioni - in particolare le esitazioni europee - ben prima degli ultimi avvenimenti. Al Consiglio affari esteri di lunedì ho osservato che avremmo dovuto aprire non solo il capitolo 22, ma avremmo dovuto aprire da tempo anche i capitoli 23 e 24 sulla giustizia e sul rispetto dei diritti fondamentali: se lo avessimo fatto, sarebbe stato il modo più efficace per influire sulla politica del Governo turco e per dare un segnale di vicinanza a quanti in Turchia manifestano per i loro diritti. Come hanno osservato alcuni commentatori turchi, per quanto sia disincantata sulle prospettive di adesione, l'opinione pubblica turca resta molto sensibile alla voce dell'Europa: la maggioranza della popolazione si sente parte del sistema europeo, soprattutto per il particolare impegno a favore dei diritti civili. La Turchia è un *partner* strategico dell'Italia. In quest'ultimo decennio le imprese italiane che operano in Turchia, con ottimi risultati, hanno raggiunto le mille unità. Operare per l'ancoraggio europeo per le riforme e per la stabilità interna del Paese è quindi essenziale anche per i nostri investimenti e per i nostri interessi economici, questo va detto apertamente e in piena trasparenza. Come ho detto, la ripresa del percorso europeo della Turchia dipenderà innanzitutto dall'evoluzione della Turchia stessa, ma la decisione di Lussemburgo è un'occasione che io mi auguro il Governo turco saprà e vorrà cogliere. Mantiene aperta una porta, ma l'esito dei negoziati è ancora tutto da scrivere, possibilmente insieme. L'Italia è sincera amica della Turchia, un Paese che io ho da sempre in modo particolare nel cuore. Ma i veri amici sono quelli che si assumono la responsabilità di parlare con franchezza anche quando le parole dette non sono gradite. Non intendiamo, come Governo italiano, vestire i panni dei moralizzatori; al contrario, vogliamo aiutare la Turchia a conciliare le sue varie anime e a riprendere con convinzione la strada delle riforme. Il mio auspicio è quindi che il Governo turco sappia accogliere il nostro appello sincero al dialogo. Allo stesso tempo, continueremo a fare di tutto perché l'Europa percorra con convinzione la strada dei negoziati di adesione, tenendo conto, come è giusto che sia, di tutti i criteri e di tutte le condizioni necessarie, ma rifuggendo da chiusure pregiudiziali.

signora Ministro, la protesta scoppiata per difendere un parco pubblico è diventata una battaglia politica per la difesa dell'identità turca, nella quale si intrecciano motivazioni religiose, sociali, politiche e generazionali, come se lo sfrenato sviluppo urbanistico, peraltro non discusso né condiviso con la popolazione, fosse la prova delle sempre maggiori mire autoritarie del Primo Ministro. Così, la tolleranza zero posta in essere da Erdogan contro giovani inermi, studenti e avvocati, ha finito col raccontare antichi rancori, e non solo l'islamismo strisciante, un paternalismo religioso soffocante, finanche il divieto di baciarsi in pubblico e di bere una birra, di dissentire da quei concetti di Patria e di islam pena il reato di blasfemia, che hanno già portato in galera decine di intellettuali; non solo, cioè, la frattura tra islamismo e laicismo, ma uno scontro più complesso. La vera posta in gioco secondo noi, signora Ministro, è la democrazia, che per Erdogan si ferma ai cittadini che l'hanno votato, dimenticando che la tutela di chi ha espresso un'opinione diversa è l'architrave decisiva sui cui si misura invece una democrazia compiuta, in cui il rapporto tra potere politico e società sia improntato sempre al valore del dialogo. Le scelte del Governo hanno esasperato le divisioni, ed Erdogan sta pericolosamente deviando verso un nuovo autoritarismo incompatibile con la libertà. Noi abbiamo in questi anni riconosciuto alcuni meriti del Primo Ministro, pur dentro ad una vicenda che ci ha visti, come lei sa, sempre esprimere solidarietà al popolo curdo. Riportare, per esempio, un Esercito con vocazioni golpiste dentro le caserme è stato un merito di Erdogan, ma a cosa è servito se poi con il tempo lui stesso si è sostituito ai militari bloccando a sua volta la la democratizzazione del Paese, e se oggi assomiglia di più ad un sultano che parla a se stesso, come se i giovani che sono per strada non fossero anch'essi figli del suo stesso popolo? L'Unione europea, forse perché un po' troppo interessata ai futuri oleodotti che probabilmente passeranno per la Turchia sottraendoci alla dipendenza dal gas della Russia, è stata incapace di svolgere un ruolo politico: e il suo silenzio è stato assordante, troppo distante da quegli Stati Uniti d'Europa che servirebbero. Il percorso di adesione della Turchia all'Unione, bloccato da dieci anni, andrebbe rilanciato - lei, Ministro, su questo ha perfettamente ragione - ma con esso anche la democrazia ed il sacro rispetto del dissenso, perché piazza Taksim non è un problema di ordine pubblico ma è un vero grido di libertà. Certo, non è la Primavera araba, ma ha con essa in comune lo stesso filo che ha attraversato le strade e le piazze in tutti questi anni: è anzitutto l'essere al di fuori della politica tradizionale, con tutti i limiti ma anche con le opportunità che questo significa. Il contagio che ha attraversato il Mediterraneo, indipendentemente se intendesse criticare efferate dittature o semplicemente democrazie sofferenti, ha avuto comunque una parola comune, pur nelle evidenti differenze che lei in questi giorni ha opportunamente sottolineato, e noi l'abbiamo condiviso. Questa parola comune è: «democrazia». Una parola, signora Ministro, che vale sempre: vale anche in quella parte del mondo che fortunatamente può votare ed esprimersi liberamente, ma nella quale, a volte, questa stessa parola allude

finestra") *(PdL)*. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, se ci avessero chiesto qualche tempo fa di fare il nome di una Nazione che fosse servita da esempio di buona *governance*, in grado di garantire pace e sicurezza, non avremmo avuto dubbi. Un esempio splendido ed inaspettato di una *governance* interna ed esterna, soprattutto nell'opera di mediazione politica internazionale in tutto il bacino mediorientale, era tutto anatolico: la Turchia. Non è un paradosso. Al cospetto della Turchia, sembrava essere proprio l'Occidente a dover imporsi una vera e radicale revisione migliorativa dei propri sistemi democratici; bastava guardare alle proteste delle piazze europee, quando ormai si sentiva impellente una rivoluzione etica che ridesse dignità alle parole, ubbidendo alle proprie Costituzioni, a cominciare da una sana cessione di sovranità. Oggi però siamo al cospetto di fatti che non rassicurano: piazza Taksim è divenuta luogo di protesta cruda e violenta, di contrapposizione al Governo che dimostra i suoi limiti, dando prova che la strada della democrazia in quel Paese è ancora lunga. Migliaia di manifestanti antigovernativi hanno chiesto a Tunali, nel centro di Ankara, le dimissioni del premier turco Erdogan. Si arrestano giornalisti ed il pugno durissimo della polizia si fa sentire. Lo scenario cui assistiamo quotidianamente è inqualificabile e pone questioni di politica internazionale serie e fondate. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, il nostro è uno Stato di diritto che ha visto digerire la democrazia di fatto negli anni che pur hanno segnato la nostra stessa storia nazionale. In quanto Stato di diritto, non possiamo che restare basiti per i fatti di cui si fa protagonista la Turchia. Non è certo un buon momento per quel Paese, ma il senso di tutto ciò che accade è gravissimo; lo si vede non tanto dai motivi del contendere, quanto da una irragionevole presa di posizione governativa, ottusa, impreparata Tutto ciò ci serve però a ridimensionare quella buona *governance* della Turchia cui accennavamo in esordio e ad adeguare, in termini di attenzione, la nostra politica estera.

cui 27 commissari hanno deciso un paio di giorni fa di riaprire la trattativa con Ankara e di portarla a compimento a partire da ottobre, nell'auspicio fortissimo - che lei ha voluto interpretare questa mattina

un processo non solo economico. Non siamo più Comunità economica europea, ma Unione europea: un'Unione che fonda i suoi principi, dopo Maastricht, su aspetti

nei programmi di studio di tipo kemalista, che erano stati attuati dopo la rivoluzione di Kemal Atatürk, a partire dal 1936, e che oggi, invece, tornano ad evidenziare purtroppo una priorità nei principi religiosi musulmani.

politica comunitaria di difesa e di organizzazione strutturata dal punto di vista militare possa diventare per questa Europa uno degli argomenti fondamentali nel prossimo futuro. Credo che anche questo possa essere un forte

Ministro, che sia giusta la sua valutazione politica, che ha riscontrato consensi e, mi pare, qualche successo diplomatico significativo: l'Europa non poteva e non doveva irrigidirsi ed alzare un muro contro muro. La questione del parco, chiamiamola la questione urbanistica della città di Istanbul, sembra sapientemente affidata ad una consultazione democratica locale. Tuttavia, le considerazioni del rapporto tra la Turchia e

Chi erano i "giovani turchi"? Nel semplicismo interpretativo si dice «liberal-massoni ufficiali formatisi nelle università di Parigi», ma erano soprattutto il frutto della diplomazia europea, del vecchio impero. Da questo punto di vista sono stati dei modernizzatori radicali non privi di qualche punta di giacobinismo, non privi di tensione (pensiamo all'eccidio armeno). Da tutto questo la Turchia è riuscita pian piano ad uscire. L'evoluzione del partito AKP è molto interessante: un partito islamico che accettava però la continuità storica della rivoluzione del 1914 e, quindi, complessivamente laico moderato. Sembrerebbe che nell'esercizio del potere questo partito stia rivelando un certo integralismo del potere. Speriamo che non sia così, ma non possiamo fare a meno di registrare i processi che ci sono stati. Lei, onorevole Ministro, ha citato intelligentemente le valutazioni di un libro di Samuel Huntington. Più concretamente, sul piano dei fatti possiamo registrare i successi e le aperture sul fronte della questione curda, una questione che poteva riesplodere a piazza Taksim. E se poi si dovesse fare un confronto, che giustamente lei ci ha suggerito di non fare, in questo momento la piazza egiziana, che sembrava foriera di primavera,

per l'Assemblea parlamentare dell'OSCE (trattasi di diplomazia dei Parlamenti, non dei Governi). L'OSCE ha deciso di svolgere i suoi lavori egualmente ad Istanbul, ma non c'è dubbio che secondo le tradizioni di civiltà democratica della nostra Assemblea ci sarà una giornata di dibattito, soprattutto per quelle violazioni dei diritti di ripresa giornalistica, e via dicendo. Credo, allora, sia molto saggia

condizioni delle carceri, materie sulle quali l'Italia non ha nessuna lezione di liberalismo e di europeismo da rivolgere all'opinione pubblica turca. turca. Non lasciamo cadere allora quell'occasione per la quale la voce dell'Europa è considerata dall'opinione pubblica turca tanto importante approviamo la decisione di recepire l'appello alla moderazione, di non irrigidirsi e di tenere aperto quello che quello che non deve più separare la Turchia dall'Europa, perché se fosse così, come parve cinque anni fa ai tempi dell'incidente con quella parte dell'Occidente che è lo Stato di Israele, se la Turchia andasse alla ricerca di ancoraggi che non fossero l'Europa e l'Occidente sarebbe una catastrofe, proprio nel senso del titolo di quel libro che denunziava, ma non auspicava, lo scontro delle civiltà. Sto citando Huntington, l'autore che anche lei, onorevole Di qui l'attenzione e la gratitudine del nostro Gruppo per le considerazioni che abbiamo avuto modo di ascoltare stamane.

piazza Taksim a Istanbul durante quest'ultimo mese è diventata non solo l'epicentro fisico della protesta di gran parte del popolo turco contro la politica di tipo «confessional-integralista» di Erdogan, ma il nuovo nucleo simbolico di un rinnovato bagliore di libertà e di un desiderio irrefrenabile di modernità culturale ed economica che sta attraversando il versante arabo del Mediterraneo già da alcuni anni. Solo la scorsa settimana eravamo qui riuniti per ratificare un documento che avrà una portata innovatrice di tipo legislativo epocale sul fondamentale tema dei diritti umani: la Convenzione di Istanbul, che ha innestato un virtuoso meccanismo di tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza; e ora, per uno strano intreccio del destino, o forse no, ci ritroviamo a discutere della Turchia proprio in senso opposto. Non come un luogo geografico dove la modernità ha trovato i suoi spazi riformatori sotto una forte spinta giuridica intrisa di democraticità nei valori e nei principi ispiratori, ma un luogo dove i diritti sostanziali stessi sono stati compressi da un vento di arcaico moralismo religioso pregno di repressione sociale, sia nei costumi sia nelle garanzie della libertà individuale universale. Chi ha avuto modo di approfondire le vicende che hanno generato la protesta dei turchi nei confronti delle scelte del Governo di Ankara si sarà accorto che siamo di fronte a una battaglia di civiltà di dimensione storica. Quella che a prima vista poteva rappresentare una contestazione che trae la sua forza dalla reazione delle nuove generazioni turche alle imposizioni legislative «moralizzanti» sugli stili di vita sollecitati dai partito filoislamico AKP di Erdogan (divieto di vendita di alcolici, riproposizione del *turban* per le donne, costruzione di nuove monumentali moschee, posizioni parlamentari omofobe) si è poi trasformata in una opposizione vigorosa alle strategie culturali ed amministrative del Paese anatolico. I giovani di Istanbul stanno rischiando da giorni la propria incolumità fisica, e purtroppo alcuni di loro sono morti, per difendere la loro dignità di Paese moderno, europeo, pienamente civile e competitivo, che ha innervato la propria struttura economica in questi anni su un sistema commerciale e finanziario di tipo capitalistico-occidentale. In sostanza, la portata rivoluzionaria della rivolta di piazza Taksim, sta nel fatto che per la prima volta un popolo islamico si sta battendo aspramente contro le scelte governative di politica amministrativa, su precise disposizioni edilizie e urbanistico-ambientali del *Premier* e del partito di maggioranza che rappresenta. Per la prima volta il monolite immutabile ed incontestabile del Corano viene messo in discussione. Per la prima volta, la supremazia «politica» della religione musulmana sugli interessi collettivi e sociali è messa sotto scacco dalla voglia di modernità culturale. Scendere per le strade e difendere dalla demolizione il parco Gezi nel cuore della millenaria odierna Istanbul, volta a far spazio a nuovi edifici religiosi e commemorativi dei passato ottomano, significa tutelare la propria identità di società occidentale evoluta e la nascita di una rinnovata coscienza civica nelle giovani generazioni. Le dure reazioni di Erdogan nei confronti delle posizioni critiche che ha giustamente espresso l'Europa sulla violenza con cui sta reprimendo la contestazione nelle varie città turche sono un segnale di debolezza del *Premier* di Ankara, il quale sembra aver perso il controllo degli eventi. Il rischio è che l'azione del Governo turco si incanali unicamente verso una pericolosa deriva di tipo soppressivo-militare. Ciò va assolutamente evitato. Per tali ragioni credo sia opportuno che il Governo italiano, per quanto sia possibile, attraverso una meticolosa ed efficiente azione di mediazione internazionale, attraverso le istituzioni a tal uopo previste dalle organizzazioni diplomatiche europee, si faccia carico di individuare soluzioni adeguate volte a contemperare e garantire tutti gli interessi contrapposti lesi e tutelare ogni diritto inviolabile calpestato. Le tensioni sociali, prima, e gli scontri di piazza, poi, pare siano figli di questa «crisi ideologica» che sta vivendo quel Paese. È sull'aspetto dei principi giuridici alla base del rispetto dei diritti umani che L'Europa può e deve fare qualcosa prima che si arrivi a una terribile guerra civile e una assurda carneficina. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli senatori, abbiamo ascoltato con attenzione l'informativa del Ministro degli affari esteri, anche se francamente, leggendo i giornali, ne avremmo potuto apprendere di più. Siamo rimasti delusi sia per il contenuto politico, che per la sfuggente azione, che per la fosca visione futura. Oggi, nella sua informativa il ministro Bonino ha riaffermato che i «turchi non sono arabi e piazza Taksim non è piazza Tahrir». E, aggiungiamo noi, non è certamente piazza San Pietro o piazza Duomo, o place de la Concord o Piccadilly Circus. Lo abbiamo sempre detto e lo ribadiamo nuovamente in questa circostanza: la Turchia non c'entra proprio nulla con l'Europa. Non c'entra culturalmente. E tanto meno storicamente. Ed è lo stesso Governo Erdogan a non riconoscere l'Europa. Anche in questa occasione le azioni della Farnesina, signora Ministro, sono state evanescenti. È così, signora Ministro, e non se ne abbia a male se diciamo la verità. Siamo anche disponibili a riconoscerle il beneficio dell'impegno, che tuttavia è annullato da una credibilità estera che l'Italia ha perso nel tempo. Non siamo più credibili in India, dove abbiamo lasciato due soldati ancora ingiustamente prigionieri. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Non lo siamo in Libia, dove il nostro brillante disimpegno a favore degli interessi delle multinazionali si è concluso con la consegna di un altro pezzo del sud Mediterraneo nelle mani dell'Islam integralista. Non lo siamo in Israele, nei cui confronti abbiamo tenuto una politica "a dente di sega". Non lo siamo più sul profilo diplomatico in generale, dopo le brutte figure del suo predecessore e di una diplomazia che - spiace dirlo - purtroppo oggi rappresenta l'ombra di quello che è stata. A proposito, quanto ci costano le nostre sgangherate rappresentanze diplomatiche all'estero? E quanto sono utili al Paese oggi? Alla persona del ministro Bonino riconosciamo schiettezza e onestà intellettuale. È per questo che da lei avremmo apprezzato che ci avesse detto le cose come stanno veramente. Qualche giorno fa il professor Sartori, commentando sul «Corriere della Sera», argomentava giudicando il Governo Letta come uno tra i più sgangherati quanto a *deficit* di competenza tra i propri Ministri. Noi non abbiamo questa opinione di lei, signora Ministro. Però le chiediamo di non farsi risucchiare dalla mediocrità delle scelte che negli ultimi anni hanno caratterizzato la politica estera italiana. Per ridare prestigio al nostro Paese non serve un politica estera imperialista, anche perché, pur volendo, il Paese non ne ha le risorse, i soldi né tanto meno la determinazione politica. Occorre invece una politica estera che sappia difendere il lavoro italiano sostenendo il commercio estero delle nostre industrie e delle nostre imprese,

tanto più alla luce di questa intollerabile svolta autoritaria con evidenti coloriture integraliste. La Turchia, non dimentichiamolo, è l'esempio di un regime che in quarant'anni ha massacrato impunemente decine di migliaia di curdi. «L'Italia vuole una Turchia pienamente democratica in Europa e l'adesione all'UE può avere un effetto benefico per la Turchia»: queste sono sue parole, signora Ministro. Ma noi non ci ritroviamo in questa sua visione. E non di certo per quanto concerne l'aspirazione di consolidamento democratico della Turchia, che tutti vogliamo, quanto piuttosto per la seconda parte della sua affermazione: non sono infatti questi i tempi per pensare a quali benefici possa avere la Turchia dall'adesione all'UE, quanto piuttosto è ora di capire che gli interessi degli italiani in Europa devono venire prima di quelli dei turchi! *(Applausi dal Gruppo Ln-Aut).* È un dato di fatto che i progressi della Turchia in termini di adeguamento ai comuni *standard* europei restano dubbi e modesti, con particolare riguardo alla parità di trattamento delle donne, al ruolo dell'esercito, al rispetto delle regole stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro. Troppo poco abbiamo trovato nelle sue parole, signora Ministro, riguardo a questi concetti. Qualsiasi ragionamento in senso inclusivo della Turchia nella UE è quindi oggi, ancor più di ieri, insostenibile. con il suo Governo musulmano-conservatore è sempre meno autorevole e sempre più autoritario ed è lo specchio della lontananza politica della Turchia dall'Europa. Alle censure giunte dalla Germania e dalla Commissione europea, Erdogan ha risposto con un duro attacco all'Europarlamento, "colpevole" di aver denunciato la feroce repressione delle manifestazioni dei giovani turchi. «Non riconosco questo Parlamento europeo», ha dichiarato Erdogan, attaccando addirittura la legittimità della prima istituzione democratica dell'Unione europea. Oggi le strade di Istanbul assomigliano più a quelle delle capitali africane arabe che a quelle di una capitale europea. Quindi, che fare? Dobbiamo affrontare la questione dei confini dell'Europa non su base geografica ma in ragione di presunte esigenze di stabilità economica o politica? No, signor Presidente, no, signora Ministro. Noi diciamo di no a questa impostazione. Portare nell'Unione europea Paesi instabili e con *deficit* di democrazia non vuol dire automaticamente renderli più democratici. E in ogni caso, prima di far entrare nella casa comune europea la Turchia, l'UE deve decidere «cosa vuol fare da grande». La politica estera del Governo in tema di allargamento dei confini dell'Unione europea assomiglia a quella politica «del ventre molle», che già si concretizza in Italia attraverso una scriteriata accoglienza di tutto e di tutti, a prescindere dalla reale sostenibilità economica, sociale e culturale delle enormi masse che premono dal sud del Mediterraneo verso i nostri confini. Negli scorsi giorni, signora Ministro, leggevo l'opinione di un noto commentatore che si interrogava sulla condotta del Governo in tema di politica estera. Oggi le rivolgerò le stesse domande. domande. Ci chiediamo, signora Ministro, come è possibile che dopo l'uccisione della cooperatrice Barbara De Anna e del capitano Giuseppe La Rosa, cinquantatreesimo militare italiano vittima del terrorismo dei talebani, l'Italia non decida di anticipare il ritiro delle proprie forze dall'Afghanistan tanto più alla luce dell'incredibile legittimazione che gli Stati Uniti hanno dato ai talebani, invitandoli a ritornare al potere dopo esserne stati scalzati nel 2001.Ha ancora senso restare in Afghanistan? Come è possibile che il Ministro degli affari esteri italiano emerga come capofila dei filoturchi in Europa, sollecitando il via libera al negoziato sull'ingresso nell'Unione europea della Turchia, proprio quando la repressione violenta delle manifestazioni pacifiche ordinata da Erdogan ha finora provocato la morte di 3 manifestanti e circa 8.000 feriti, mentre altre 11 persone hanno perso la vita e 59 versano in gravi condizioni? Queste domande nascono dalla reale sensazione che la politica estera italiana oggi non conti nulla e che il Governo non sia affatto «sul pezzo» e che stia invece impegnando la residua credibilità del Paese in scelte anacronistiche e sfasate rispetto alla realtà, come dimostra l'atteggiamento di rinnovata considerazione per l'adesione della Turchia all'Unione europea. No, signora Ministro, non ci stiamo! La sua stringata informativa conferma che la politica estera italiana continua a rimanere marginale e inadeguata rispetto a una pluralità di problematiche, a partire dalla necessità di affermare chiaramente in sede europea che occorre porre un termine preciso all'insostenibile politica di allargamento dei confini dell'Unione europea

In conclusione, signora Ministro, in tema di priorità le ribadiamo: cosa aspettiamo a riportare a casa i nostri soldati dall'Afghanistan? Mancano le risorse per i servizi sociali principali nei Comuni e l'Italia continua a spendere miliardi di euro per partecipare, peraltro in maniera totalmente subalterna, ad operazioni militari estere che hanno perso di significato anche per i nostri principali alleati. Assistiamo da troppi anni ad annunci di ritiro mentre si continuano invece a rifinanziare missioni estere ormai inutili,

Si abbia piuttosto la dignità di porre fine a questo sacrificio di risorse e di vite. Una volta ogni tanto, facciamo noi una scelta nel nostro interesse, per primi, senza agire, come al solito, in maniera subalterna agli altri *partner* internazionali.

sottolineo: giustamente - é partita dal Governo Berlusconi. E io credo che su Berlusconi e sulla sua politica estera si possano esprimere tanti giudizi, ma sulla Turchia condivido pienamente quello che è stato un investimento di fiducia di quel Governo rivolto con preveggenza al futuro. Cari colleghi, negli anni successivi ai Governi Berlusconi ci sono stati Governi del centrosinistra che non hanno modificato l'impostazione verso la Turchia. E oggi il Ministro degli affari esteri è venuto in piena continuità con quelle politiche che (almeno una volta diciamocelo tra noi) sono state un minimo comune denominatore positivo della politica estera italiana. Infatti, potete aver detto anche cose giuste, perché tutti noi siamo inorriditi dal fatto che Erdogan disconosca la legittimità del Parlamento europeo e lo attacchi nel modo volgare in cui lo ha attaccato; tutti noi riteniamo inaccettabile la repressione dei diritti legittimi dei manifestanti. tutti noi dobbiamo porci una domanda, che è quella decisiva nella politica estera del nostro e degli altri Paesi: chiudere quella porta significa ottenere più sicurezza, più Europa, significa salvaguardare gli interessi dell'Occidente, dell'Europa, dell'Italia, o significa fare un atto straordinario di autolesionismo politico? È un atto straordinario di autolesionismo politico. E io sono ben contento che il Ministro abbia

avviso, è questa: i veri amici parlano chiaro. Noi siamo veri amici della Turchia, lo abbiamo dimostrato con una continuità di politica governativa in questi anni, e, proprio perché siamo veri amici, dobbiamo parlare chiaro

Turchia, che, con tutti i limiti del caso, anzitutto è una democrazia: si svolgono le elezioni, si vince e si perde. Scusatemi, ma vista l'area politica in cui è situata la Turchia, francamente non mi sembra che sia un particolare del tutto indifferente. luogo, la Turchia è nella NATO: sappiamo di che cosa stiamo parlando, sappiamo che cosa significa la presenza della Turchia nella NATO. In terzo luogo,

Infine, la Turchia è un *partner* commerciale importantissimo per le aziende, per gli imprenditori italiani, per l'economia italiana. È chiaro che quella di queste ore è anche una crisi di crescita, una crisi di benessere; c'è un'esplosione del ceto medio che fino a vent'anni fa era un essere indefinito, cioè non esisteva in Turchia, e questo confligge con un'impostazione tradizionalista dal punto di vista religioso. Nel merito ci sarebbero tante riflessioni da fare: il benessere e il rapporto con la religione, questioni molto interessanti (ma forse sarebbe bene in quel caso fare un seminario, più che trattarle in questo dibattito così rapido).

i turchi sono contenti perché non vogliono che andiamo a sindacare adesso, aprendo questo capitolo, su quello che è stato l'inaccettabile metodo che il Governo ha usato nel reprimere;

della contentezza sono esattamente opposte, ma questo rinvio, in fin dei conti, è stato l'atto più intelligente che si poteva fare, perché da parte nostra significa dire ai turchi che se continuano così non ci va bene quello che sta capitando è inaccettabile rispetto ai nostri *standard*, e puruttavia loro restano artefici del loro destino: noi non chiudiamo loro le porte, non lo facciamo oggi perché sarebbe un errore.

su questi capitoli. Onorevoli colleghi, piazza Taksim non è piazza Tahrir: ha detto bene il ministro Bonino e ha fatto bene a ripeterlo, perché è ingiusta una semplificazione di questo tipo. Poi voi dite che non è neanche piazza San Pietro; sì, non è piazza San Pietro, non è piazza Duomo e non è piazza Maggiore di Bologna, ma questo lo sappiamo tutti. Qui siamo a Istanbul: conosciamo la storia,

In conclusione, noi siamo con il Governo e per la continuità di questa politica estera. Naturalmente, il capitolo che lascio all'immaginazione dei presenti è che sono convinto e sicuro che quando il Ministro degli affari esteri si siederà con le autorità turche, poiché ha un sentimento di grande attenzione alla Turchia (che personalmente condivido e del quale sono partecipe), da vera amica saprà spiegare tutte le cose che non ci vanno bene (e sono tante).

la Turchia è un grande Paese. La Repubblica turca creata da Kemal Atatürk sta

Ci sono altri aspetti che vorrei ricordare, che rendono sicuramente questo Paese un *partner* estremamente importante per l'Italia e per l'Europa. La sua posizione strategica ne ha fatto un importante membro della NATO. La sua natura euroasiatica ha determinato questo lungo e non ancora compiuto negoziato per l'ingresso nell'Unione europea: un negoziato travagliato al punto tale che la Turchia ha chiesto e ottenuto di entrare anche nella *Shanghai* *Cooperation Organization*. Quindi, non una linea come quella prima detta dal collega della Lega Nord, ma una linea completamente diversa e molto più significativa per noi e per la politica estera estera dell'Unione europea, perché ha aperto una linea di intesa ad Est del tutto inedita e ha mostrato, con le parole del ministro degli affari esteri Davutoglu, che la Turchia può garantirsi dei margini di manovra autonomi nella propria collocazione nello scacchiere internazionale. La Turchia ha coltivato una relazione privilegiata con i Paesi turcofoni dell'ex Unione Sovietica, che sono un elemento importante nelle politiche energetiche. Ha coltivato anche una relazione privilegiata con i Paesi musulmani, soprattutto quelli di lingua araba, dove negli ultimi trent'anni sono state intensificate, con la fondazione di scuole, fondazione di scuole, queste relazioni culturali. È stato intensificato uno scambio, che sicuramente potrebbe tornare importante anche per le politiche del Mediterraneo che sicuramente ha determinato una grande crescita economica anche nella penisola anatolica. Un elemento fondamentale per noi - per l'Italia, per l'Europa e per le nostre relazioni con la Turchia

per uno slittamento verso una islamizzazione, prima ancora dell'economia, più che della società. Dunque, la Turchia è un *partner* importante, ma anche molto delicato. Per questo vorrei tornare un momento su un aspetto che è collegato all'annuncio fatto di aprire in ottobre il Capitolo 22. è stato dato in un momento particolarmente caldo, sia per la mancanza di dialogo tra Erdogan e lo scontro aperto tra la popolazione e i suoi rappresentanti, sia per delle fratture che ha aperto all'interno dell'AKP (il partito di governo, di Erdogan) e per le dichiarazioni sprezzanti che Erdogan ha avuto nei confronti della reprimenda ricevuta dal Parlamento europeo per le violenze contro i manifestanti e le parole dure e intransigenti. Allora noi, come il presidente Casini, ci domandiamo: che senso diamo a questo annuncio? senso diamo a questo annuncio? Si è voluto avallare la politica di Erdogan, proprio nel momento in cui è stato contestato più massicciamente dall'inizio della sua carriera politica, avallando in qualche modo la sua presa di posizione antidemocratica? si è voluto dare, come si suggeriva poc'anzi, una sorta di *warning*, stabilendo quindi un periodo di osservazione delle sue prossime mosse? Oppure ancora, semplicemente, si teme che la durata negli anni e la difficoltà nella manovra di avvicinamento tra Unione europea e Turchia abbiano definitivamente spinto la Turchia a orientarsi verso linee diverse e ad allearsi con altri soggetti internazionali? O cosa forse ancora più grave per l'Unione europea - si teme che questo periodo di prova, di qui ad a ottobre, significhi che ancora una volta, a distanza di meno di un mese

Certo, una Turchia stabile e democratica avrebbe un ruolo importante per affrontare temi nevralgici per l'Europa e per l'intero Mediterraneo: commercio, energia, ambiente, migrazioni, ma anche sicurezza e prevenzione dei conflitti. potrebbe essere un sostegno al processo di democratizzazione dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. La sua laicità potrebbe costituire un forte segnale contro la tendenza - che ho sentito anche nelle parole dei colleghi - di rappresentare i conflitti in Medio Oriente come uno scontro di civiltà tra Occidente e mondo musulmano, nascondendone così, sotto questo pretesto, le cause vere, spesso legate ad interessi economici e non certo a differenze culturali

del fatto che i valori su cui si basa una prospettiva futura dell'Europa non hanno corrispondenza in credenze religiose ma le superano, possono prescinderne, possono andare avanti e possono essere il rispetto dei diritti dell'uomo, a prescindere da questo. L'ingresso della Turchia nell'Unione europea si profila sicuramente come portatore di grandi cambiamenti, non solo economici ma anche per la stessa identità.

portata ad assumere un ruolo di grande responsabilità nelle politiche del Mediterraneo, che potrebbe effettivamente sinergicamente condividere con una Turchia europea? Signora Ministro, sappiamo che la credibilità nella politica estera dipende dalla credibilità di quello che va molto di moda chiamare «sistema Paese», quindi è giocoforza che il quesito si sposti: signora Ministro, non ritiene che sia indispensabile pretendere che nel Consiglio dei ministri, di cui lei fa parte, si perseguano con forza e non a parole quelle politiche che rendono un Paese più credibile agli occhi della comunità internazionale? Mi riferisco ad una seria e produttiva lotta alla corruzione, corruzione, all'evasione e all'elusione fiscale, alla promozione della ricerca e della cultura, alla valorizzazione delle eccellenze, al sostegno e all'affermazione dei diritti e della libertà di informazione. Quanto ai recenti fatti di violenza perpetrati dalle forze di polizia turche contro i manifestanti, mi preme sottolineare che quella dimostrazione è nata da un *sit-in* in piazza Taksim, nel cuore della parte europea più giovane e moderna, laica proiettata verso la dimensione internazionale di quella incredibile città sospesa tra due continenti. Una dimostrazione in difesa di un parco, ma in realtà in difesa di una città che uno sfrenato sviluppo urbanistico vorrebbe modificare, per meglio dire plasmare, senza risparmiare quartieri storici simbolo della Turchia kemalista del secolo scorso, come Nisantasi, Osman Bey, Haydarpasa solo per fare qualche nome. Una reazione, finalmente, allo sfrenato desiderio di lasciare un segno, di trasformare dei luoghi nel riflesso di un diverso sistema di valori, in cui la volgare patacca di un centro commerciale travestito da finta caserma ottomana incontra la voglia di consumo di un Paese in enorme crescita economica e paradossalmente si accompagna con il sempre più diffuso divieto di bere alcool. segni, esempi della linea politica che sempre più vuole dare il primo ministro Erdogan, che proprio qui, come sindaco di questa città, ha iniziato a mostrare insofferenza per la sostanza laica della Costituzione. La sua politica in questa occasione in tutta la sua dimensione autoritaria, determinata a imporre valori e stile di vita conservatori al resto della società turca. Così la risposta è finalmente arrivata. Queste voci sono state inascoltate da Erdogan con arroganza e, anzi, fronteggiate con una violenza inaudita, e questo è stato fatto in ordine a precise sue indicazioni, il che ha provocato l'esplosione della tensione, smentendo e annullando i tentativi di un atteggiamento conciliante del presidente Gül e perfino del vice primo ministro Arinç.

l'intervento del presidente Casini, che sicuramente ha dato un quadro assolutamente condivisibile. Occorre premettere che la Turchia è da decenni un *partner* strategico dello schieramento occidentale, nel suo insostituibile ruolo di cerniera tra Europa e Asia.

basati su un laicismo illuminato, sono stati affermati da Kemal Atatürk all'indomani della caduta dell'Impero Ottomano. Negli ultimi anni inoltre la Turchia ha goduto di stabilità e crescita economica assolutamente straordinarie e molte sono le nostre imprese che vi hanno costituito

e che dovevano essere superati di slancio i veti e le riserve di tanta parte dell'opinione pubblica nordeuropea e anche italiana. Era e rimane troppo importante, sotto il profilo strategico, economico, geopolitico e anche culturale, tenere legato allo schieramento occidentale questo straordinario Paese. Chi parla pertanto può considerarsi a tutti gli effetti un amico della Turchia. Ciò detto, è tuttavia innegabile che la Turchia negli ultimi anni ha subito, al pari di molti Paesi della sponda sud del Mediterraneo, una pericolosa regressione e involuzione. Il Partito per la giustizia e lo sviluppo di governo del *premier* Erdogan, al potere da oltre dieci anni, che si dichiara islamico moderato, ha in verità ripudiato l'illuminata eredità di Kemal Atatürk e ha favorito una reislamizzazione delle istituzioni turche: esempio, alla reintroduzione del velo per le donne negli uffici pubblici, ma vi sono altri aspetti che sono stati ricordati in quest'Aula. Persecuzioni e discriminazioni culturali ha subito anche la minoranza cristiana in questi anni. A questo arretramento culturale e civile, ad un autoritarismo nazionalista hanno reagito le frange più giovani e culturalmente più evolute della società turca, che hanno dato vita alle manifestazioni di piazza Taksim, a Istanbul, e nelle principali città. Abbiamo assistito sgomenti ad una violenta repressione di queste manifestazioni. Va, quindi, denunciato in questa sede, senza se e senza ma, l'uso irragionevole e sproporzionato della forza da parte del Governo turco nei confronti dei manifestanti. Tutta la mia umana e politica solidarietà va ai giovani rimasti ciechi per i gas lacrimogeni urticanti, alle centinaia o migliaia di feriti, ai colleghi avvocati arrestati per essersi messi a disposizione degli incarcerati. Questi sono eccessi che vanno stigmatizzati e denunciati con la massima fermezza. E questo può farlo l'Italia, signora Ministro, con l'autorevolezza che deriva dal fatto di essere da sempre Nazione amica della Turchia, con rapporti bilaterali particolarmente cordiali e fecondi, sviluppati anche negli anni recenti del Governo Berlusconi, come ricordato Una volta tanto, signora Ministro, possiamo davvero dire, a buona ragione, che il nostro ruolo ci consente di svolgere un'azione di mediazione e di stimolo al dialogo democratico, con maggiore credibilità ed efficacia rispetto ad altri Paesi, magari anche economicamente più forti di noi. Certamente - bisogna ahimè riconoscerlo - l'atteggiamento sfrontato del presidente Erdogan non aiuta a distendere l'atmosfera. Per tutta risposta ad una risoluzione comune del Parlamento europeo, che condannava la repressione violenta delle manifestazioni, Erdogan ha affermato di non riconoscere alcuna decisione presa dall'Europarlamento sulla Turchia. Tra l'altro, la risoluzione che era stata approvata era abbastanza blanda e si limitava ad esprimere preoccupazione per l'uso sproporzionato della forza e a manifestare timori per il deterioramento della libertà di stampa. Ciò detto, in modo chiaro e netto, occorre a mio giudizio ribadire che rimaniamo amici e alleati della Turchia. Bene ha fatto quindi il nostro Paese a favorire la riapertura ad ottobre del negoziato per la sua adesione all'Unione europea. In questo quadro, la Turchia dovrà essere aiutata a tutelare meglio i diritti civili e le minoranze religiose. Ma guai ad isolarla, spingendola verso l'islamismo e l'estremismo! Questo davvero non possiamo permetterlo. Dopo gli errori di valutazione che lo schieramento occidentale ha commesso in Libia e in Egitto e che rischia ancora di commettere in Siria, Paesi dove le cosiddette primavere arabe hanno prodotto solo caos, anarchia e violenza, dove oggi i nostri fratelli cristiani e i ceti borghesi ormai rimpiangono senza esitazioni l'*ancien régime* e dove gli unici a esultare sono i salafiti ed i jihadisti, occorre riconoscere che solo il dialogo e il negoziato portano buoni frutti, non gli strappi e le accelerazioni dei processi politici. La stabilità del quadrante sud del Mediterraneo passa inevitabilmente attraverso un ruolo forte della Turchia, che deve continuare a trovare nel nostro Paese e nell'Unione europea dei *partner* stabili ed affidabili, garanti al contempo di democrazia e sviluppo economico.

Gli americani direbbero: *thank you for your leadership*. È un vero esempio di *leadership* la linea che grazie a lei il Governo italiano ha assunto in questo passaggio così delicato e così difficile; è stato un atto di *leadership* dire nei giorni scorsi, anche sfidando la impopolarità del momento, che piazza Taksim non è piazza Tahrir, ma resta un fatto vero e giusto, ed è quindi giusto dirlo, anche perché sentiamo tutti il bisogno, nella politica in generale e nella politica estera in modo particolare, di punti di riferimento chiari e di lungo periodo. Non si può fare politica in generale e politica estera in modo particolare senza stelle fisse, senza punti di riferimento chiari, altrimenti si finisce per sbandare emotivamente, prendendo anche colossali granchi e quindi facendo disastri sul piano politico nazionale e ancor più internazionale. Ciò non significa che la politica in generale e anche quella estera non debba lasciarsi attraversare dalle emozioni. Tutti abbiamo provato forti emozioni nel vedere le immagini di piazza Taksim: sentimento di riprovazione, di condanna, di sdegno nei confronti dei gravi abusi della forza che sono stati perpetrati, e che non possiamo che condannare con grande fermezza,

da scolpire: la democrazia non è solo vincere le elezioni, ma è innanzitutto, prima ancora delle elezioni, rispetto per le minoranze. Ci sono tante dittature che hanno vinto le elezioni, ma non c'è nessuna dittatura che rispetti le minoranze. La differenza tra dittatura e democrazia è il rispetto delle minoranze. *(Applausi Il punto politico resta quello che lei ha detto e che noi condividiamo pienamente, cioè che questi rischi di involuzione della Turchia non a caso si si sono verificati in coincidenza con l'impallidire della prospettiva di integrazione della Turchia in Europa. Vale quindi anche il rovescio: l'unico modo per dare struttura e prospettiva chiara, certa e affidabile ad un percorso di evoluzione democratica e liberale della Turchia non può che essere quello di rilanciare la prospettiva europea. Per questo motivo, ringrazio il nostro Governo e in particolare la ministra Bonino, che si è battuta con grande determinazione in sede europea per riaprire questa porta. Mi si consenta di dire che vale anche il reciproco.

della politica estera comune a livello europeo. Quando attuiamo la politica intergovernativa e andiamo in ordine sparso, facciamo grandi figuracce a livello internazionale, quando l'Europa riesce a parlare con una prospettiva chiara e unitaria produce grandi risultati. Pensiamo ai risultati storici raggiunti nei Balcani.

Paesi che sono stati teatro di massacri e che oggi hanno, appunto, la prospettiva dell'ingresso in Europa. Mi viene anche da dire che, quando abbiamo smesso di guardare alla Turchia con interesse, con attenzione, con generosità e apertura,

nazionale. Solo quando si apre e sa proporre al mondo la sua prospettiva unificante, l'Europa è forte ed è capace anche di produrre risultati in altri terreni, come quelli decisivi e strategici dell'unione economica.

Si potrà discutere sulle primogeniture (non credo che Romano Prodi abbia imparato da Berlusconi la crucialità della Turchia, ma al riguardo ognuno ha le proprie ricostruzioni), tuttavia l'aspetto fondamentale è che questa politica verso la Turchia, di fermezza e di apertura al tempo stesso, è l'elemento unificante del nostro Parlamento ed è, in questo momento, un punto chiave della politica estera del Governo. Pensiamo che questo possa restare a lungo uno dei punti chiave di una politica estera comune e anche di quel bipolarismo convergente che auspichiamo torni ad essere il punto di snodo del nostro sistema politico quando questa fase avrà raggiunto, come il presidente Napolitano auspica continuamente, i suoi risultati di rafforzamento della nostra prospettiva democratica.

Signora Presidente, intervengo per esprimere la solidarietà del Movimento 5 Stelle al sindaco di Pomezia Fabio Fucci, al vice sindaco Elisabetta Serra e al vigile urbano che nella giornata di ieri sono stati aggrediti a calci e pugni nella piazza di quella città da quelli che i *media* hanno definito venditori ambulanti insoddisfatti dalla negata autorizzazione per l'allestimento di un mercato a Torvaianica. Peccato che uno degli aggressori, tale Walter Fedele, sia stato anche sindaco della stessa città negli anni Novanta, quindi ben consapevole del ruolo e della responsabilità di un primo cittadino. Noi, come in ogni occasione, condanniamo decisamente la violenza, nei confronti di chiunque venga esercitata, ma non siamo convinti che in questa occasione tale violenza sia semplicemente frutto dell'esasperazione nei confronti di un rappresentante delle istituzioni (rappresentante che, è bene ricordarlo, ha assunto tale carica la prima volta in assoluto circa dieci giorni fa e che precedentemente era esponente della minoranza). Noi temiamo si tratti di un vero e proprio atto intimidatorio, nei confronti di un esponente del Movimento che già in passato ha ricevuto minacce da un consigliere di altra parte politica. Ribadiamo dunque la solidarietà e la vicinanza alle persone vittime di questo episodio increscioso e chiediamo alle autorità competenti di fare piena luce sull'intera vicenda.

ore 20,58, la torre di controllo di Ciampino perde le tracce del DC9 Itavia, con a bordo 77 passeggeri, di cui - se non ricordo male - dieci bambini e quattro membri dell'equipaggio.

L'aereo era partito da Bologna ed era in volo verso la Sicilia. Dopo 33 anni i familiari delle vittime e noi tutti cittadini attendiamo ancora di veder cadere la cortina d'omertà e di vedere rischiararsi l'opacità e sparire le ombre che ancora pesano insopportabilmente su questa tragedia ed ostacolano il raggiungimento della verità. Certo, non sempre si può arrivare a verità, ma sempre si deve rispettare la tensione alla verità, poiché pensiamo che, in un Paese come l'Italia, che si professa democratico e civile, sempre si debba lottare per la conquista della verità. Ciò non è altro che una lotta per ottenere e tutelare il diritto alla giustizia. Nel commemorare la strage di Ustica, noi del Movimento 5 Stelle desideriamo ricordare una ad una le 81 vittime, pregando i colleghi di alzarsi e di ascoltare in silenzio i nomi, non solo in segno di rispetto, ma anche come assunzione di una responsabilità: quella di fare tutto ciò che è necessario per assicurare giustizia e verità. E ora leggo ad uno ad uno i nomi di queste 81 persone, perché a ciascuno di loro corrisponde una famiglia, una famiglia che ancora sta aspettando giustizia e verità.

come l'aereo è caduto per una bomba collocata a bordo e come tutte le ricostruzioni di fantascienza, che hanno imbrogliato l'immaginario collettivo - la battaglia aerea, il missile - sono solo nella testa dei giornalisti che si sono arricchiti attraverso questi libri di fantascienza. Se vogliamo parlare della verità,

la ricorrenza così drammatica della strage di Ustica. Com'è noto, su questa strage ci sono tante ipotesi, che hanno animato anche un dibattito molto acceso nel corso di questi anni. Tuttavia, siamo di fronte ad uno dei grandi misteri non gloriosi del nostro Paese. È un mistero che ne accompagna altri e l'elenco sarebbe lungo quasi quanto quello delle vittime della strage di Ustica, partendo dalla strage di piazza Fontana e a seguire.

certe cose si facciano con il preavviso necessario e con un coinvolgimento dell'Aula, come deve essere), che sulla strage di Ustica la Presidenza, magari non nell'immediato, ma in un momento successivo, ci consenta di svolgere un confronto, un dibattito che parta dal riconoscimento di questa giusta

Signora Presidente, innanzitutto vorrei ricordare che questa mattina ho appreso dai *media* che colui il quale rappresenta l'unità nazionale, cioè il Presidente della Repubblica, ha inviato un messaggio ai familiari delle vittime, auspicando che sia fatta chiarezza. Ciò significa che il nostro Presidente riconosce che qualcosa di non chiaro c'è, ed il Presidente della Repubblica ci rappresenta tutti.

Presidente, comprendiamo bene l'imbarazzo che prova la Presidenza di fronte a certe situazioni.

Signora Presidente, mi rammarico dell'equivoco verificatosi, perché il nostro responsabile d'Aula, nel segnalare il mio intervento di fine seduta, si è anche premurato di segnalare il contenuto dell'intervento. Ci dispiace, pertanto, e ci rammarichiamo che ci venga imputata la colpa di una mancanza di tempismo grave, della Presidenza, che non ha tempestivamente ricordato e commemorato questa strage che andava ricordata e commemorata all'inizio della seduta.

La seduta è ripresa.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalla mattina di martedì 2 luglio, alle ore 11, per l'esame del decreto‑legge in materia di efficienza energetica e misure fiscali nonché per la discussione congiunta del disegno di legge di delegazione europea 2013, della Legge europea 2013 e delle connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Saranno inoltre esaminate ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione esteri. Nel corso delle discussioni generali dei provvedimenti citati 1a Commissione permanente è autorizzata a riunirsi per l'esame del disegno di legge costituzionale recante l'istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali. Per quanto riguarda la settimana successiva alla prossima, con inizio dal pomeriggio di lunedì 8 luglio, il calendario prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, l'esame del predetto disegno di legge costituzionale. Saranno inoltre discusse le mozioni sulla partecipazione dell'Italia al progetto dell'aereo militare F35, nonché il decreto-legge sull'IMU e gli ammortizzatori sociali, approvato alla Camera dei deputati, ove concluso dalle Commissioni. La seduta è tolta